L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

dei colleghi De Castro, Di Nardo, Andria, Pertoldi, Santini, Fontana, Bertuzzi, Pinzger, Montani, Mongiello e Piccioni, quasi tutti membri della Commissione agricoltura e produzione agroalimentare del Senato che so con quanta passione e con quanta onestà intellettuale hanno seguito questo provvedimento fin dall'inizio e continuano a seguire tutte le questioni che riguardano l'agricoltura italiana di cui si occupa ogni giorno il Governo e, in particolare, il ministro Luca Zaia. Dispiace avere notato in alcuni interventi

un po' ingeneroso non tanto nei confronti di chi vi parla, che non ha bisogno di alcun tipo di generosità da parte di alcuno,

cercando di offrire al Ministro un contributo emendativo migliorativo. Devo dire che da parte del Ministro c'è stata, sinora, una buona capacità di ascolto. Non è del tutto esatta, colleghi, nemmeno l'affermazione secondo la quale non vi sarebbe stato alcun tipo di ascolto nei confronti dell'opposizione o delle opposizioni: anche se

come emendamenti co-firmati dai senatori del Popolo della Libertà, della Lega Nord, del Partito Democratico e dell'Italia dei Valori, cioè dell'intera Assemblea. Non mi sembra, quindi, del tutto esatto quanto è stato detto. Vi

polemica che è logico accettare nella discussione di un provvedimento di questo tipo - nel fare un richiamo continuo all'onestà: vorrei fosse chiaro, colleghi, signor Ministro,

non ci sia bisogno di ricordare tutti gli emendamenti che sono stati approvati in Commissione, in quanto ne abbiamo parlato diffusamente questa mattina e ne riparlerà, se lo riterrà, il Ministro più tardi.

all'inizio ha avuto difficoltà ad accettare questa impostazione, ma poi è venuto incontro con intelligenza alla pressione forte che è arrivata in particolare dal Gruppo del Popolo della Libertà, della Libertà, cui ha dato ragione, ribaltando in questo modo un contenuto non secondario del decreto originario.

euro. Vi renderete conto, colleghi, che qualcuno di voi ha chiesto qualcosa di oggettivamente fuori dalla realtà. È vero che il Ministro aveva dichiarato che vi sarebbero stati questi 500 milioni di euro, ma a tale cifra si arriva attraverso 35 milioni di euro, che speriamo possano essere approvati come previsto da un emendamento, che moltiplicati per 10 attraverso il moltiplicatore, visto che ora stiamo parlando di un fondo di garanzia, più il 50 per cento di cofinanziamento vanno a garantire un importo pari sostanzialmente più che coperto quanto previsto e promesso dal Ministro in una delle sue precedenti dichiarazioni. Colleghi, credo occorra procedere come abbiamo fatto finora, presto, bene e prendendo in considerazione

il suo *iter* in quanto andrà alla Camera dei deputati dove potrà essere ulteriormente migliorato. Credo che i nostri colleghi della Camera dei deputati avranno modo di dimostrare il proprio valore

ad un provvedimento ulteriormente migliorato e tuttora perfettibile. Credo che da parte del Governo vi sia la necessaria capacità di ascolto, la stessa capacità che ha cercato di dimostrare, spero riuscendovi, il relatore in questo ramo del Parlamento. Parlamento. Abbiamo ancora qualche settimana per un lavoro successivo alla Camera, che potrà conferire al provvedimento in esame, ne sono certo, quella dignità che in questo momento molti rappresentanti dell'opposizione non gli Per quanto riguarda il variegato mondo agricolo italiano, alcuni hanno ritenuto di fare un lavoro sottotraccia, emendativo, concreto, ora per ora, dialogando con il Ministro e con me per portare a casa un provvedimento accettabile, buono e capace di evitare all'Italia di pagare, il prossimo anno, 170 milioni di euro di multa sul latte - perché di questo stiamo parlando

difficile e quotidiano che abbiamo portato avanti insieme a lei in questi giorni, in Commissione agricoltura del Senato, ci permette oggi di guardare a questo provvedimento

Sono presenti in tribuna, per una visita al Senato, gli studenti dell'Istituto comprensivo «Vincenzo Scamozzi» di Vicenza. A loro e ai loro insegnanti indirizziamo il nostro saluto e gli auguri per la loro attività di studio.

ho ascoltato con attenzione tutte le dichiarazioni relative al decreto-legge in esame. Prima di entrare nel merito di una valutazione molto compiuta e spero anche puntuale

che ha accompagnato il provvedimento, i parlamentari della maggioranza e dell'opposizione e tutti i lavoratori e dipendenti del Ministero che hanno contribuito alla redazione di questo provvedimento.

fu chiuso in modo opportuno in Europa. Forse quella notte qualcuno si è distratto, e l'Italia ne è uscita con una quota latte pari a metà del suo fabbisogno. Ancora oggi, su 20 milioni di tonnellate di latte che si consumano in Italia, 10.800.000 sono prodotte dalle nostre 40.000 stalle, sono prodotte dalle nostre 40.000 stalle, ma l'altra quantità, oltre 10 milioni di tonnellate, viene importata da altri Paesi. Abbiamo chiuso un negoziato sfortunato, che ha significato per lo Stato membro Italia un pagamento di 3 miliardi di multe, a tutt'oggi, che ha pesato nei negoziati che abbiamo tessuto e intrattenuto in Europa in questi anni per circa 9 miliardi di euro.

ovvio che, di fronte alla possibilità di dar corso a operazioni esecutive, quindi di messa all'asta delle aziende, e alla riscossione forzosa forzosa delle multe, abbiamo deciso che si potesse dare un'ulteriore opportunità a queste 8.404 aziende. Da qui nasce l'idea di questo negoziato con l'Europa - che con l'Europa abbiamo voluto condividere giorno dopo giorno - che ci permette di proporre a

distribuendo la quota a queste tre categorie, quindi attribuendo quote latte a chi già produce e ha bisogno di entrare nell'alveo della legalità con le proprie produzioni, e avendo riconosciuto, nel caso di affittuari e di quota B, le proprie produzioni. Il secondo: nessuna

di una rateizzazione in totale regime di aiuti di Stato con interessi zero. Oggi parliamo di una rateizzazione, come dicevo prima, molto più importante e molto più onerosa.

1. 1. È convertito in legge il decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4, recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. BONFRISCO, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo, con le seguenti condizioni rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che all'articolo 2, al comma 2, siano aggiunte in fine le seguenti parole: "Alla istituzione e alla tenuta del Registro di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente"; che all'articolo 4, al comma 5, siano soppresse le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2011 sulle competenze di cui al presente comma provvede l'AGEA"; che all'articolo 4, dopo il comma 2, sia inserito il seguente: "2-*bis*. i produttori devono esprimere la rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari". In ordine agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.13, 1.402, 3.401, 4.1, 4.2, 4.3, 4.3, 4.6, 4.7, 4.8, 4.13, 4.0.200, 4.22, 4.23, 6.1, 6.2, 6.5, 6.6, 6.10, 6.0.1, 6.0.200, 6.0.201, 6.0.300, 6.400, 6.700, 6.10/1, 6.10/2 e 6.10/3. Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 4.33. Esprime parere non ostativo su tutte le restanti proposte, ad eccezione che sull'emendamento 6.0.5 sul quale il parere è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione, al capoverso 4, dell'ultimo periodo».

che ci è stata fornita dal Ministero dell'economia e delle finanze, regolarmente bollinata dal Ragioniere generale dello Stato, soltanto poche ore fa. Molto rapidamente, signor Presidente, vorrei illustrarle di cosa si tratta. In una prima Nota tecnica di integrazione della Relazione tecnica, anch'essa regolarmente bollinata dal Ragioniere, il Ministero dell'economia scriveva (questa è la Nota tecnica del 17 febbraio) che, in merito agli effetti finanziari in termini di fabbisogno derivanti dalla prescritta rateizzazione, si ritiene in primo luogo - attenzione, signor Presidente - che si possa presumere la neutralità dell'iniziativa (è evidente che si sta parlando della neutralità finanziaria), in considerazione del fatto che l'interesse attivo sulle somme da rateizzare risulta di fatto superiore al tasso di approvvigionamento delle somme sul mercato.

io Stato devo incassare dei soldi da un privato; se il privato non mi paga (un privato obbligato a pagarmi), io Stato gli consento una rateizzazione e lo faccio, o meglio - consentitemi di dirlo - pretendo di farlo, senza un onere in capo al bilancio pubblico (nemmeno un onere di cassa, se non di competenza), perché l'interesse che faccio pagare al privato in questione è uguale, o addirittura superiore, a quello pagato in quel momento sui titoli di Stato a medio termine. Signor Presidente, non è difficile capire cosa succederebbe del bilancio pubblico se si procedesse in questo modo con chiunque abbia debiti da pagare allo Stato. In pratica, non ci sarebbe più nessun privato che pagherebbe regolarmente perché tutti chiederebbero la rateizzazione e lo Stato sarebbe costretto a consentirla semplicemente imponendo il pagamento di un tasso di interesse uguale a quello in quel momento praticato sui titoli di Stato a medio termine. Sulla base della valutazione circa l'assoluta incongruità della tesi in rapporto alla legge di contabilità - e mi consenta, signor Presidente, anche in rapporto al buonsenso

Proprio oggi pomeriggio, è arrivata una nuova Nota integrativa del Ministero dell'economia, anche questa regolarmente bollinata dal Ragioniere generale dello Stato,

Infatti, scrive il Ministero dell'economia: «Al riguardo si fa presente che, nel caso in esame», cioè quello di questo provvedimento e di questa rateizzazione, «anche in considerazione dell'andamento del fabbisogno tendenziale e sulla base delle risultanze dell'attività di monitoraggio, nelle previsioni tendenziali dei saldi di finanza pubblica, non si è tenuto conto» - attenzione, non si è tenuto conto -«prudenzialmente degli effetti derivanti dal recupero delle somme dovute dai produttori del settore lattiero‑caseario. Tali debiti sono da sempre risultati, infatti, scarsamente onorati». Ho letto esattamente il contenuto dell'integrazione della Relazione tecnica. non ha mai segnalato, nei mesi e negli anni scorsi - mi sto riferendo, quindi, ad un periodo di tempo molto lungo - al momento del calcolo del tendenziale, per esempio in termini di fabbisogno, che si stava determinando un grave scostamento rispetto alla legislazione vigente nell'andamento delle entrate derivanti dall'applicazione della legislazione vigente stessa in materia di quote latte.

«Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative.».

la questione ha una sua complessità tecnica, ma, insisto, mi riferisco alla Presidenza del Senato e a lei, che sta presiedendo in questo momento l'Aula, perché, in realtà, la questione che voglio porre ha uno squisito significato istituzionale. Non mi sto riferendo, di conseguenza, al Governo. Il Ministro dell'economia, signor Presidente, in materia di attuazione della legislazione vigente sulle quote latte insisto - non ha fatto uso dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge n. 468; un articolo che obbliga il Governo, ove si determini uno scostamento in termini di entrata e in termini di spesa, in fase di attuazione della legislazione vigente, a segnalare il fatto al Parlamento, in modo che il Parlamento possa adottare le conseguenti misure di ripiano della scopertura che si sta determinando in sede di attuazione della legislazione vigente stessa.

ci dice che non ha tenuto conto, al momento in cui ha calcolato il tendenziale nel bilancio a legislazione vigente sul versante del fabbisogno, delle entrate relative

dell'applicazione della legislazione vigente in materia di quote latte. Signor Presidente, vorrei che avessimo chiaro tutti il fatto che stiamo parlando di 1.300.000.000 di euro

stante il bilancio a legislazione vigente, che copre la legislazione vigente, se il Parlamento fa un'innovazione legislativa di tipo oneroso deve disporre, per rispettare l'articolo 81 della Costituzione, le risorse necessarie per fare fronte all'onere determinato dall'innovazione legislativa stessa. Signor Presidente, vorrei fosse chiaro che, su questa base e sulla base della Nota oggi inviataci, il Ministero dell'economia cancella l'articolo 81 della Costituzione e, soprattutto, soprattutto, rende vana la nozione stessa di copertura finanziaria alla luce dell'articolo 81 della Costituzione. È molto facile dimostrarlo, perché basta porre qualche domanda.

sotto il profilo del fabbisogno si vorrà segnalare al Parlamento che si sta determinando uno scostamento di tali dimensioni, tra le entrate previste a legislazione vigente e quelle che, di fatto, si prevede possano essere effettivamente realizzate, incidendo di conseguenza sulla cassa e quindi anche sul fabbisogno?

Noi stiamo ponendo una domanda molto semplice: questo è l'unico caso in cui il bilancio a legislazione vigente è stato fatto, senza segnalare il problema al Parlamento, in termini difformi rispetto a quanto previsto dalla stessa legislazione vigente? È questo l'unico caso o ce ne sono degli altri? Se ce ne sono degli altri, quali sono?

E io non credo che si possa procedere all'esame degli articoli di questo disegno di legge prima che a questa domanda sia stata data una risposta convincente. Faccio notare, signor Presidente, che, a dimostrazione del fatto che quello che dico almeno qualche fondamento ce l'ha (secondo me, più d'uno),

ma, signor Presidente, così pone un problema di carattere istituzionale enorme. Qual è la sede del potere di decisione sul bilancio? È il Parlamento, come stabilisce la Costituzione, oppure

evidente, signor Presidente, che si sta ponendo una questione di portata istituzionale assolutamente di prima grandezza. *(Applausi dai Gruppi PD e

Innanzitutto, le questioni si ponevano su due livelli: una con riguardo ai flussi, cioè al modo in cui viene regolato il versamento di questo debito nei confronti dello Stato

è stato attentamente analizzato come, a fronte di una rateizzazione delle entrate e di un interesse su tale rateizzazione, si è approvvigionato lo Stato con una provvista che, addirittura, costa un po' meno dell'interesse che pagano i debitori nei confronti dello Stato. È assicurato, dunque, che sul piano dei flussi viene rispettata la correttezza della tenuta dei conti pubblici.

è stato correttamente compilato, quindi non si pone un problema in termini di competenza e dunque d'indebitamento netto. nella critica anche dei documenti che sono stati presentati alla Commissione bilancio, si deve considerare che non si è costruito un bilancio che non teneva conto di questo grande credito dello Stato nei confronti di alcuni produttori, ma ci si deve riferire soltanto al conto di Tesoreria dello stesso. Il conto di Tesoreria - lo ricordo solo a me stesso - attiene esclusivamente al fabbisogno e quindi, di seguito, di seguito, al debito dello Stato; sostanzialmente, è una sola partita finanziaria che, come ho detto prima, non incide sulla competenza economica e quindi sul bilancio dello Stato propriamente detto. la questione delle anticipazioni di Tesoreria, la Relazione tecnica del provvedimento innanzitutto già pone la questione (da lì si è acceso il faro sulla Commissione bilancio) ed indica con correttezza che questa partita è stata regolata, in lunghi anni e con tutti i Governi che si sono succeduti, come mera partita finanziaria, quindi un'anticipazione di tesoreria ed un conto di tesoreria che è stato lì appostato. È vero che, all'entrata del conto di tesoreria, non è stata appostata alcuna somma, ma su questo mi soffermerò tra un momento. quanto alla legislazione vigente, sulla parte in conto capitale, è ormai da tempo, come si sostiene nella nota della Ragioneria generale presentataci, che il tendenziale di bilancio viene assunto come parametro di quantificazione, come dimostrano peraltro le varie relazioni tecniche alla legge finanziaria. Questo significa che il parere di osservanza dell'articolo 81 è stato correttamente espresso dalla Commissione, perché perché se il tendenziale viene assunto come parametro di quantificazione, la Nota della Ragioneria ha detto correttamente che non è stato modificato il tendenziale in maniera difforme da quella prevista e da quella necessaria. Sul piano sostanziale - questo osservo al senatore Morando - credo essendo stato vittima di una questione del genere in altra legislatura, su un altro problema riguardante in quel caso l'agricoltura, tutto sommato bene abbia fatto chi ha visto quel conto di tesoreria a non ascrivere in entrata somme che si sapeva non sarebbero state versate. Se fosse un bilancio civilistico - mi rendo conto che non è questo il caso, ma vale la pena di fare un ragionamento analogico - direi che quel parametro è stato costruito in maniera prudenziale. Si è detto «Che cosa scrivo in entrata se sono ragionevolmente certo che non ci sono entrate?» E così è stato. Per questa ragione è evidente che quella valutazione è stata prudenziale. Se ai fini del parametro "legge di contabilità" si possono fare alcune osservazioni, se al fine della discrezionalità di una simile valutazione si possono fare delle osservazioni, è certo però che quel parametro è stato

sulla costruzione del bilancio a legislazione vigente e se, come credo, questa discussione sarà utile farla anche in sede di dibattito di una riforma del bilancio, penso che quella sarà la sede per affinare gli strumenti di comunicazione al Parlamento su alcune vicende particolari che riguardano il bilancio dello Stato. in più. Concludendo, affermo che correttamente, ai sensi della legislazione vigente, il parere è stato dato dalla Commissione bilancio senza il riferimento all'inosservanza dell'articolo 81. Sul piano formale alcune questioni si sono poste anche questa volta, ma era avvenuto anche in altre materie, e correttamente ci si porrà il problema nella sede propria che è la Commissione bilancio. Sul piano sostanziale possiamo dire che il bilancio si ritrova

credo che le argomentazioni del senatore Morando dovrebbero convincere noi tutti dell'opportunità (ripeto: soprattutto dell'opportunità) di sospendere l'esame del provvedimento che abbiamo davanti. È fin È fin troppo evidente, infatti, che stiamo affrontando una questione di straordinaria delicatezza, che non è nell'interesse di nessuno, tanto meno di una delle due Camere, affrontare come un tema di importanza minore da posporre ad un momento successivo. Se quelle argomentazioni non fossero sufficienti, proverò a "rifrasarle" in maniera leggermente diversa. Ho molto apprezzato la misura straordinaria del Ministro delle politiche agricole e anche del relatore del provvedimento, i quali si sono sforzati di suggerire che questo provvedimento non comporta oneri per lo Stato e addirittura evita alcune spese. In realtà, sono stati molto modesti, perché a leggere bene la Nota della Ragioneria generale dello Stato questo provvedimento fa emergere risorse e determina un miglioramento del fabbisogno;

di non poter prendere provvedimenti importanti perché ha a cuore le sorti del nostro debito, la soluzione ce l'ha davanti: un paio di provvedimenti di questo genere e possiamo tranquillamente finanziare la riforma degli ammortizzatori sociali, e non solo, forse potremmo spingerci anche più in là. Ma non basta. Questo provvedimento, se lo prendete per un attimo sul serio, schiude prospettive straordinarie anche per affrontare la crisi. Pensateci un attimo: alla luce della nota della Ragioneria Generale dello Stato, diventa incomprensibile il comportamento delle banche che sostengono, a volte, che allungare le scadenze per loro è costoso; infatti, se è vera la Nota della Ragioneria Generale dello Stato, allungare le scadenze ottiene l'effetto di far emergere risorse e non di imporre un onere al creditore. Vorrei sottolineare al presidente Azzollini che, se fossimo di fronte ad un bilancio civilistico, non è affatto vero che prudenzialmente dimenticheremmo un'entrata; in realtà, quello che faremmo sarebbe appostare una sopravvenienza passiva (e la vedremmo chiaramente in bilancio) oppure costruire una riserva a fronte di un'entrata poco certa. Ciò che è accaduto qui è invece qualcosa di assai più serio, ossia la discrezionale omissione di una voce di entrata che, è vero, ha effetti sul fabbisogno, ma cela in realtà al Parlamento la dimensione dei problemi economici che si trova ad affrontare. Guardate, non è un problema di poca rilevanza. Capisco che il Ministro dell'economia abbia detto più volte che bisogna superare le attuali regole contabili, ma stiamo andando troppo oltre rispetto al voluto e al necessario. È evidente che, se le cose vengono affrontate come questa nota ci dice, stiamo svuotando di ogni significato

un atto di rispetto nei confronti di un organismo come la Ragioneria generale dello Stato, che non è e non vuole essere il luogo dell'opacità, ma credo che sia e voglia essere il luogo della trasparenza, nell'interesse del Parlamento e del Paese.

bilancio. La fretta a volte può essere cattiva consigliera e mi riferisco, presidente Azzollini, all'ultimo parere che venne espresso, in fretta,

agli enti previdenziali degli immobili invenduti, che erano anche soggetti a contenzioso, operazione priva della copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, come era stato rilevato in quest'Aula dai colleghi del Partito Democratico.

quel parere emanato in fretta dalla Commissione bilancio del Senato ha trovato le critiche da parte della Commissione bilancio della Camera.

ad essere più rigorosi nei criteri di trasparenza del bilancio dello Stato.

Ho ascoltato con grande attenzione le argomentazioni del senatore Morando e del senatore Rossi e prendo atto di quanto da loro dichiarato. dell'Aula, non tanto il problema specifico delle quote latte, nella tecnicalità che è già stata illustrata dal presidente Azzollini, piuttosto, una situazione istituzionalmente grave, nella quale il Parlamento decide del bilancio dello Stato e della legge finanziaria

che ben due leggi finanziarie del Governo Prodi si sono basate esattamente su questo trucco contabile:

il trucco? Sta nel lasciare la definizione di legislazione vigente alla discrezionalità della Ragioneria generale dello Stato; e allora basta abbassare l'andamento tendenziale delle entrate per poi, in tempi successivi, gridare: «Ohibò, ohibò, abbiamo fatto la lotta all'evasione: le entrate sono maggiori e quindi ci sono miliardi e miliardi di tesoretti!». Non era un problema di maggioranza e opposizione allora, non è un problema di maggioranza e opposizione oggi: è un problema istituzionale, per mettere il Parlamento in condizione di avere un numero di partenza che sia certificato e trasparente, e quindi un'autorità indipendente che riferisca su questo alle Camere. Questo è il compito che, tra l'altro, la Commissione finanze ha già intrapreso sulla base della relazione della Corte dei conti, che ha già indicato cifre ballerine, proprio per questi criteri, che oscillano tra i 20 e i 30 miliardi. Sono quindi favorevole a procedere su questo specifico disegno di legge, ma mi asterrò dal

ma all'aderenza dell'agire del Governo e del Parlamento all'articolo 81 della Costituzione e alla legge sulla contabilità pubblica. di altro che di questo. E il fatto che la cifra, come dice il presidente Azzollini, sia contenuta, non sposta di un millimetro la questione. Noi abbiamo già avanzato la richiesta, che rinnoviamo, sperando che sia onorata, per non dover aggiungere un altro elemento di straordinaria difficoltà nelle relazioni tra maggioranza, Governo e opposizione a quelle che già esistono e che riguardano una certa disinvoltura nell'osservanza delle regole costituzionali ogni qual volta il Governo si trova a presentare un provvedimento in quest'Aula, troppo spesso un decreto-legge: noi chiediamo che il ministro Tremonti venga in Senato e risponda all'obiezione che abbiamo posto con molta serietà

rilevanza e delicatezza da porlo di fronte alla più alte cariche dello Stato. Mi auguro che da parte dei rappresentanti del Governo, che certamente colgono la delicatezza della questione, questa richiesta venga accolta. Considereremmo molto grave il fatto che venisse disattesa. finestra"). Come ho già detto, informerò il presidente Schifani e valuteremo questa richiesta al Governo. Del resto, mi sembra che il dibattito, al di là della differenza di comportamento e di voto

di chi, essendo in regola con i versamenti delle multe, ha diritto ad eventuali restituzioni di quote che dovessero risultassero in eccesso. È conseguentemente necessario sopprimere il comma 4-*quater* attraverso cui il Governo intende alimentare il fondo a sostegno del settore latteario-caseario con eventuali restituzioni di quote in eccesso. Noi riteniamo questo un fondo importantissimo, ma che dev'essere alimentato con gli interessi delle rate dei "supersplafonatori" e non a danno di chi le rate le ha sempre pagate.

D'altra parte, trovo importante anche il ragionamento fatto dal Ministro e soprattutto l'accoglimento

al Ministro per l'accoglimento dell'emendamento 1.35 che va a favore della zootecnia di montagna.

l'emendamento 1.26 che intende stabilire un ordine di priorità nelle assegnazioni in modo da evitare che siano gli splafonatori ad essere avvantaggiati rispetto agli affittuari che hanno osservato il rispetto delle regole. Per questa ragione, si chiede con questo emendamento che le assegnazioni siano destinate in primo luogo alle aziende che hanno subìto la riduzione della quota B; in secondo luogo alle aziende ubicate in zone di pianura e svantaggiate che, nel periodo 2007-2008, risultano produttori affittuari di quota; ed infine ad aziende che abbiano prodotto oltre la propria quota, ovvero i cosiddetti splafonatori.

*(PD)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, illustro il subemendamento 1.401/1,

alla definizione del procedimento di rateizzazione. Ritengo questa una proposta indispensabile ed opportuna proprio per assicurare l'effettivo pagamento delle multe prima dell'assegnazione delle quote e al tempo stesso non ostacolare la partenza del percorso di assegnazione delle nuove quote. Vorrei sottoporre all'Assemblea, signora Presidente, due aspetti fondamentali della questione: uno riguarda il fatto che le quote devono essere assegnate in riserva nazionale prima e non dopo le adesioni degli splafonatori; nello stesso tempo, le assegnazioni devono riguardare tutti i produttori con prelievo non versato. Ritengo questo un emendamento opportuno e indispensabile, come dicevo prima, per non mortificare i tanti allevatori onesti che nel corso di questi anni hanno pagato le quote, talvolta indebitandosi, e mettendo a rischio, in alcuni momenti, la sopravvivenza delle loro stesse aziende.

anzi doveva illustrarli tutti, visto che ha avuto la parola. Può intervenire in dichiarazione di voto, senatore Andria.

1.401 (testo 2).

del debito e soprattutto a ridimensionare la durata dello stesso. Quindi, l'intenzione emendativa è quella di riportare ad una durata massima di 20 anni il periodo della rateizzazione. in modo da indicare esplicitamente che la durata della rateizzazione non superi i tre anni quando il debito è inferiore ai 10.000 euro, non superi i dieci anni per i debiti inferiori ai 100.000 euro e non superi i 20 anni per i debiti superiori ai 100.000 euro.

ripristinare una dimensione del fondo più congrua rispetto ai fabbisogni di quelle aziende che hanno regolarmente acquisito le quote sottoponendosi ad importanti investimenti. Pertanto, il passaggio da 25 milioni a 100 milioni consente di ripristinare molto più velocemente l'importo minimo necessario a supportare le aziende che nel corso di questi anni hanno tenuto un comportamento regolare

si intende far affluire le somme versate dai produttori di latte in un conto di tesoreria destinato all'estinzione delle anticipazioni a favore dell'Agenzia dovute alla mancata riscossione dei crediti del settore agricolo. Inoltre, la differenza tra interessi applicati e rendimenti dei buoni del Tesoro potrà essere riassegnata al Ministero delle politiche agricole per interventi nel settore lattiero-caseario e per operazioni di ristrutturazione del debito e di accesso al credito per gli operatori del settore. Dunque, l'intenzione che è alla base di questo emendamento è quella di

più volte nel corso del dibattito in Commissione agricoltura e che riguardano evidentemente argomenti di estrema delicatezza ed importanza, perché gli agricoltori queste misure le hanno regolarmente ottenute negli anni precedenti. quello di cui ci stiamo occupando, in sostanza, è il mantenimento di ciò che è stato garantito dal precedente Governo nella precedente legislatura. Questo riguarda sia la proroga previdenziale sia il Fondo di solidarietà nazionale. Ci rimettiamo, evidentemente, al parere che la Commissione bilancio ha dato, ma la speranza è che si riesca a dare oggi una risposta sia all'uno sia all'altro

che fa propria la sostanza dell'emendamento precedente della Commissione, portando la proroga delle agevolazioni contributive fino al 31 dicembre di quest'anno.

e così drammatico per il potere d'acquisto delle famiglie italiane, che ogni giorno si trovano sempre più in difficoltà a far quadrare il bilancio familiare, in una fase dove già sono stati persi centinaia di migliaia di posti di lavoro con altri lavoratori a rischio senza neppure gli ammortizzatori sociali, l'operazione di scontare ulteriormente prezzi già scontati, oltre ad apparire assurda, è stata un *boomerang*, uno scivolone che poteva essere evitato. Termino il mio intervento, signora Presidente, auspicando che